sabato 13 novembre a Rangoon in Birmania è stata liberata una donna coraggiosa, Aung San Suu Kyi,

lei, auspicandone la liberazione, oltre alla difesa dei diritti umani in quel Paese. Sono certa che in questo momento il nostro applauso è

quelli che purtroppo non sono ancora stati liberati. Sono tante le vittime di quei regimi odiosi che perseguitano la libertà dall'errore. Il PdL è sempre stato custode dei valori della libertà dell'errore. Con questi sentimenti, accediamo pienamente allo spirito della richiesta avanzata dalla senatrice Soliani. Signor Presidente, anche da parte del Gruppo della Lega Nord volevamo esprimere ed associarci alle parole della senatrice Soliani per quanto è avvenuto in Birmania. è una terra in cui - ahimè! - tante volte i diritti umani sono stati calpestati. Ed è anche una terra dove diversi missionari, senatrice Soliani, già dal secolo scorso hanno cominciato un'opera di ricostruzione sociale di quel popolo così martoriato. Tra l'altro, anche da Lecco, la mia città, mia città, è andato un celebre missionario a fondare centri per la cura dei lebbrosi. Per noi è questa l'occasione per ribadire la soddisfazione per tale evento e per ricordare che al mondo occorre lavorare molto per far sì che le persone che vengono così

democrazia sia riconosciuta a seguito di questa liberazione. So che nel Paese c'è molta fibrillazione in questo momento

di questo tipo che vi sono nel mondo, ovvero che quella ostinazione buona che c'è stata nel volere segnalare questo stato di sofferenza si è poi rivelata utile per la persona e credo anche per tutti quelli che alla libertà guardano come un segno ed un modello irrinunciabile per questa civiltà.

affinché i praticanti possano svolgere un tirocinio professionale adeguato e retribuito. Nel momento in cui si pone come limite all'attività di chi vuole affacciarsi alla libera professione l'incompatibilità con il lavoro pubblico o con il lavoro privato, anche *part time*, è evidente

la pratica legale: se il tirocinante non verrà pagato adeguatamente dallo studio legale (oltre tutto, avete anche stabilito che dovrà essere pagato al secondo anno della sua presenza presso lo studio),

siccome sono molto desideroso di apprendere dei profili regolamentari, vorrei capire qual è la *ratio* di una preclusione che viene dichiarata su un emendamento che, su uno stesso problema, propone una soluzione diversa ed alternativa a quella prevista dall'emendamento la cui bocciatura avrebbe determinato una preclusione. Francamente, non riesco a comprendere.

propone un compenso commisurato alla tariffa vigente nella misura minima ridotta della metà.

individua una soluzione a questo problema. Tale soluzione, signor Presidente, signori relatori, a noi sembra assolutamente inadeguata. Soprattutto, a mio modo di vedere, ove approvata, costituirà fonte di contenzioso e di problemi interpretativi di notevole rilievo. L'emendamento della Commissione, che proponiamo di integrare con il subemendamento

«commisurato» - questo è il criterio valutativo del rimborso forfetario ovvero del compenso forfetario che spetterebbe al praticante avvocato - «all'effettivo apporto dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio». Ogni studio legale italiano,

Credo sia una norma (chiedo scusa, signor relatore, non so chi l'ha proposta: non c'è nulla di irriverente ed offensivo nelle cose che sto dicendo) molto pasticciata, di di difficilissima applicazione, che sarà fonte di problemi nei rapporti tra i giovani e il *dominus* dello studio, considerando anche il il carattere chiaramente subordinato - in senso sostanziale, non in termini di rapporto di lavoro subordinato - del giovane nei confronti del suo *dominus*, che deve insegnargli ad esercitare la professione e così via. Se vogliamo dare una soluzione a questo problema, che è un problema molto serio, decidiamo una cosa che si capisca, signor Presidente e signor relatore, quale che essa sia, relatore, quale che essa sia, perché questo problema, oltre ad affrontare un tema, quello della remunerazione di un'attività lavorativa (peraltro dal secondo anno dall'avvio della pratica forense), a mio modo di vedere può contribuire a risolvere anche il tema del numero dei giovani che accedono alla professione. È del tutto evidente che se uno studio legale dovrà riconoscere un compenso, seppur minimo, ai giovani praticanti, l'avvocato rifletterà prima di dire sì ad un giovane praticante e probabilmente gli dirà sì se è un giovane di valore, se è un giovane che effettivamente vuole fare l'avvocato e quindi vuole avviare questa attività di praticantato, quando sappiamo perfettamente che oggi l'attività di praticantato è una sorta di parcheggio in attesa che il giovane trovi una soluzione lavorativa o un altro sbocco professionale. Quindi, la soluzione che io propongo (naturalmente può essere rivista, discussa o sistemata come riteniamo) è di individuare un criterio chiaro di determinazione del compenso minimo, un criterio minimale: si prevede che l'apporto del giovane venga remunerato sulla base del minimo tariffario (e sappiamo che il minimo tariffario è una misura generalmente molto bassa) ridotto della metà. A me sembra una soglia accettabile, un criterio comprensibile, che dà certezza ai giovani praticanti e agli studi che decidono

il relatore a cambiare posizione sull'emendamento stesso.

il motivo ispiratore di tutte le nostre proposte è stato quello di guardare ai giovani, prima di tutto. Ne abbiamo parlato con il relatore e con la maggioranza: prima sebbene, per il primo anno non venga attribuita nessuna ricompensa, dal primo anno in avanti si prevede un compenso forfetario. Mi rendo conto delle spese di studio di un avvocato ma, quantomeno, si garantisca un minimo, quel minimo previsto dal Consiglio dell'ordine. Appare veramente incredibile che,

**Il Senato non approva.**

come ha rilevato poco fa il collega Legnini, in questo testo noi qualifichiamo, in un primo tempo, ciò che viene erogato al praticante con il termine «rimborso». Subito dopo, però chiariamo che questo «rimborso» non è tale, ma è retribuzione, è corrispettivo per l'opera prestata:

cassiamo una sentenza relativa ai locali occupati attualmente dal Consiglio nazionale forense presso l'Amministrazione della giustizia, cosa del tutto impropria,

pattuito. Il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato, presso gli uffici legali delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici nonché presso gli uffici giudiziari deve essere svolto a titolo gratuito.». **39.252** [LI

*b)* si riferisce alle ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età,

Per questo credo valga la pena almeno di riformulare la lettera *c)* del comma 11 dell'articolo 39. gli interventi del senatore Ichino sono sempre molto pungenti. In questo caso, l'arma è fortemente spuntata, perché egli fa dire alla norma una cosa diversa da quella che effettivamente dispone. Il Consiglio nazionale forense ha il diritto-dovere di fissare i limiti

necessari e sufficienti perché quel tirocinio valga anche in Italia. Vorremo evitare, professor Ichino, che i nostri giovani pieni di buona volontà

la pratica forense non si faccia o non si possa fare o non si debba fare negli altri Paesi europei. Bisognerebbe, infatti, incidere sulla normativa europea per far sì che vi sia una legislazione uniforme a livello comunitario.

regola nell'attività professionale. L'idea che ci possa essere una preclusione o una limitazione rispetto alla formazione professionale fatta

votazione. Siccome gli altri 26 Stati membri dell'Unione europea non hanno ancora adottato una normativa stringente come la nostra, cosa succederebbe se un cittadino italiano dovesse andare a fare il tirocinio in uno studio dovesse andare a fare il tirocinio in uno studio legale americano con sede a Londra, visto e considerato che noi riconosciamo tutta una serie di

con questa norma non escludiamo la possibilità per un praticante italiano di fare uno o due anni di tirocinio in uno studio statunitense con sede in un altro Stato dell'Unione europea. Per questo mi asterrò. [LI

Ciò che si doveva scrivere - e che penso si volesse scrivere - era che il Consiglio nazionale forense disciplina con regolamento i requisiti di validità

la possibilità di cambiare il luogo in cui intende proseguire il tirocinio, dando al Consiglio dell'ordine la possibilità di autorizzare il trasferimento:

«Al praticante sarà concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputerà necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure» (per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio). Crediamo utile che sia

un regime clerico-fascista, abbiamo legalizzato il divorzio. In questo caso, invece, ci deve essere l'indissolubilità del rapporto tra il tirocinante e lo studio legale: per analogia, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di non limitare la libertà di scelta.

Si fa così perché c'è la ripresa diretta televisiva su Internet: io ogni tanto l'ho fatto. Molti lo fanno! Fate finta di non sapere che una cosa è il trasferimento da uno studio all'altro all'interno dello

39 merita una motivazione precisa, perché l'articolo ha per oggetto una questione importante e delicata. Questa motivazione poi varrà anche come introduzione alla discussione sui sei articoli successivi.

e professionale dalla vecchia generazione alla nuova, è il momento in cui un giovane traduce 16-18 anni di formazione scolastica e universitaria in competenza professionale, è il momento in cui la crisalide diventa farfalla. La questione, però, è delicata perché la proporzione tra le prestazioni oggetto del rapporto (la prestazione lavorativa del praticante e la prestazione formativa dell'avvocato dell'avvocato maturo) è una proporzione non riconducibile a standard, è una proporzione che varia da rapporto a rapporto, da caso a caso, ma anche nell'ambito del singolo caso. All'inizio il praticante sovente assorbe dal professionista una quantità di energia formativa molto superiore rispetto all'utilità che il praticante stesso dà allo studio; se le cose vanno come devono andare, il rapporto si inverte, e il professionista maturo trae dal lavoro del praticante una lauta ricompensa formativo iniziale. Tutto questo è difficile da ricondurre a uno standard e ci pone, come legislatori, un problema di difficile soluzione: per un verso dobbiamo evitare che lo stabilire degli standard minimi di trattamento finisca col deprimere l'offerta di opportunità di formazione e di tirocinio ai giovani. Questo evidentemente è un primo problema che dobbiamo risolvere. Ma c'è anche il problema

un panorama di esperienze legislative o regolamentari ricco di indicazioni. Nel Regno Unito, ad esempio, c'è un regolamento interessante che disciplina questa materia, come

il problema previdenziale, il problema di chi non riuscendo a superare il praticantato vira verso occupazioni diverse in gestioni previdenziali diverse, o viceversa chi arriva al praticantato avendo accumulato un periodo di contribuzione previdenziale in altra gestione diversa da quella della cassa avvocati. Regno Unito, dopo tre mesi di praticantato, il tirocinante ha diritto ad un compenso minimo

Ora, non dico che possiamo trasferire meccanicamente questi standard nel nostro Paese, anche perché, dobbiamo riconoscerlo, i giovani che escono da una *law* *school* britannica sono molto meglio formati di quelli che escono dalle nostre università; però, colleghi, vi chiedo: quando il tirocinio si è svolto per tutto un primo anno, se le cose si sono svolte in modo corretto e regolare,

che, almeno dall'inizio del secondo anno di pratica, ai nostri giovani praticanti si riconosca il diritto a un minimo di retribuzione. Non vogliamo adottare la tecnica proposta dal collega Legnini di una percentuale della tariffa minima relativa alle pratiche seguite dai praticanti? Possiamo allora

italiano. Vi è poi la previdenza. Vogliamo porci il problema della ricongiunzione, della totalizzazione dei periodi contributivi nei casi frequenti in cui il giovane passa da una gestione previdenziale all'altra?

che imponeva addirittura uno sbarramento per l'accesso al tirocinio; ma per il resto, da queste disposizioni che stiamo per votare

perché è compenso per l'attività svolta. Qui confessiamo la simulazione, confessiamo una gherminella verbale con cui vogliamo impedire al fisco di compiere il suo prelievo sul compenso erogato. voi a sostenere che le tariffe minime sono necessarie per garantire la dignità della prestazione forense, e ciò in riferimento ad un rapporto, quello tra tra l'avvocato e il suo cliente, che non soffre di nessuna delle distorsioni che sono invece tipiche nel rapporto che si instaura con un giovane che entra per la prima volta nel mercato del lavoro.

Voteremo dunque contro questo articolo, perché in esso si compendiano tutti i caratteri di una legge che sostanzialmente è scritta dagli *insider* contro gli *outsider*.

di corporativismo della normativa su cui stiamo discutendo, per cercare di darle un tono più moderno, più europeo, più modulato sulla prospettiva di formare

in particolare delle competenze di tipo paranormativo di questo organismo di rappresentanza degli avvocati. La norma, così come è concepita nel disegno di legge, attribuisce al Consiglio nazionale forense la potestà di disciplinare in generale,

all'esito dell'acquisizione di apporti conoscitivi, tecnici, scientifici e professionali delle diverse categorie, rispetto alle quali trasversalmente si pone la questione della formazione dei giovani avvocati. Per rendere più comprensibile ciò che ho appena cercato di spiegare, sottolineo che il comma 2 del nostro articolo, integralmente sostitutivo di quello contenuto nel disegno di legge, precisa che il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Consiglio nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, ed acquisito il parere del CSM nonché del CNEL, adotta i regolamenti

si occupa di disciplina dal punto di vista normativo e giudicante, e definisce i termini di una formazione che richiederebbe apporti da diversi soggetti, così come noi suggeriamo. Questo è uno dei punti qualificanti dell'articolo che proponiamo in sostituzione di

effettuato frequentando corsi di formazione a contenuto professionalizzante. La norma di cui all'articolo 41 contenuta nel disegno di legge allude a una frequenza obbligatoria per un periodo non inferiore a 24 mesi, laddove una prospettiva di corretta flessibilità, nell'ordine di idee cui abbiamo ripetutamente fatto riferimento di una formazione articolata, variegata e modulare suggerisce l'indicazione del diverso termine indicato nel comma

successione delle operazioni parlamentari si è commesso l'errore di richiamare testualmente ciò che è contenuto nella lettera *b)* dell'articolo 41 del disegno di legge, e in particolare, purtroppo, una parola che nel nostro vocabolario non esiste, inserita, con ironica capacità di accostamento, vicino vicino all'indicazione della necessità di insegnare il linguaggio giuridico ai giovani avvocati. Si prevede infatti che è necessario «l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti». Mi dolgo di non aver letto con adeguata attenzione, perché il termine «impugnatoria» nel vocabolario della lingua italiana non esiste.

A questo punto inizia un'opera che altro non può definirsi che di riduzione del danno. In particolar modo, i nostri

professione di avvocato)* 1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati

Noi prevediamo poi anche l'incentivazione della proposta di questi corsi e specifichiamo che «dovranno essere incentivati corsi di formazione di durata maggiore, che permetteranno, per ogni mese di corso frequentato, di abbreviare di un mese la pratica da svolgersi presso lo studio professionale». Qui potrebbe, appunto, risiedere la novità, nel senso che prevediamo pure una durata maggiore ma, in qualche modo, riduciamo la durata della pratica

di persone che hanno conseguito la laurea e che, in qualche modo, svolgono la pratica presso uno studio. Evitiamo che questi diventino avvocati quando, più o meno, saranno nell'età della pensione. Se allunghiamo troppo i tempi essi non entreranno mai nel mondo del lavoro, ma continueranno ad essere studenti o praticanti forse per troppo tempo.

obbligatoria per un periodo non inferiore a 24 mesi, ma poi si attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di fissare la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a 160 ore.

francamente troppo esoso nei confronti del praticante, il quale, dopo due anni, deve poter accedere all'esame di Stato per lo svolgimento della professione. L'obbligo dei corsi

ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a che alla lettera *a)* siano soppresse le parole "e tendenzialmentea

insistono e si impegnano affinché questa riforma vada avanti. Qual è il motivo dell'urgenza di questa riforma? Va rivista non solo perché la normativa attuale è vecchia di decenni, ma perché abbiamo nel Paese un numero rilevantissimo di iscritti all'ordine degli avvocati, avvocati, e c'è un numero non irrilevante di essi che non sono adeguati: cioè, l'inadeguatezza professionale di un numero non minimale ma piuttosto rilevante impone di rivedere l'organizzazione e la struttura di questo momento essenziale dell'amministrazione della giustizia.

che le cose vadano in maniera decisamente migliore. Ecco allora che è il momento della formazione che dovrebbe vederci più attenti e semmai più uniti. stato detto in precedenza da alcuni colleghi dell'errore grave che si commette affidando al Consiglio nazionale forense il compito esclusivo di fare tutto. tutto. È una chiusura che dal punto di vista culturale non è adeguata ai tempi e dal punto di vista strutturale non garantisce l'adeguata formazione professionale, l'organizzazione di questo momento così delicato. Pertanto, con la nostra proposta non affidiamo certo a qualsiasi altro soggetto che non sia il Consiglio nazionale forense, ma al Ministro

i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, la Conferenza dei presidi delle facoltà

con il quale ci stiamo misurando della questione economica e quindi dell'improcedibilità o inammissibilità di alcuni emendamenti. Non avete voluto - non ne comprendo le ragioni - che l'università assolvesse a un compito più elevato e -

"tendenzialmente a carattere gratuito" sarebbe stato finalmente un vero riconoscimento dei diritti fondamentali che sono parte della nostra Costituzione. non la gratuità ma tendenzialmente un aiuto a quella parte di giovani che, pur avendo grandi capacità, si vedranno ancora una volta selezionati, e quindi esclusi, sulla base di una differenza di censo.

all'arbitrio o alla scelta, che potrebbe diventare non confacente all'esigenza di un livello che ci auguriamo sempre più alto ed adeguato dell'avvocatura per il sistema giustizia. L'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale - ricordo in questa sede le battaglie

pregiudiziale o stragiudiziale - e la tecnica di ricerca sono in sostanza quelle caratteristiche che non possono mancare nella figura dell'avvocato moderno, del legale del terzo millennio. Le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato, nonché quelle per la verifica finale del profitto dovrebbero essere affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari in modo da garantire l'omogeneità di giudizio su tutto le ragioni per le quali si è contrari ad una formulazione che contribuirebbe a migliorare e a dare maggiori risultati ad una legge che, sia pure in modo piuttosto contrastato tra maggioranza e opposizione, sta andando avanti. Dette considerazioni - secondo me - dovrebbero far riflettere la maggioranza e far quindi accettare l'emendamento che ho testé commentato.

L'onorevole collega Maritati, mentre leggeva l'emendamento 41.208, ha saltato uno degli elementi più affascinanti di detta proposta,

acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario, che non è assolutamente previsto, né direttamente né indirettamente, nello stesso emendamento ai punti *a)*, *b)* e *c)*. e *c)*. In realtà una fonte culturale rispettabilissima tenta di dare al CSM, ogni volta che se ne presenta l'occasione, e anche quando non ce ne dovrebbe essere, ancora più potere

«L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 41 prevede che il Consiglio nazionale forense possa istituire verifiche intermedie e finali del profitto nell'ambito dei corsi di formazione. Ciò significa che il Consiglio nazionale forense può introdurre una serie illimitata di sbarramenti e di ulteriori esami nel corso dell'erogazione di quella formazione cosiddetta frontale, che avviene attraverso i corsi cui fa riferimento l'articolo 41.

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: «Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

stiamo formulando pareri, stiamo votando per dare al Paese leggi nuove. L'aspettativa del Paese è che finalmente cessi questo atteggiamento. Qui non si tratta di dare più potere al Consiglio superiore della magistratura ma di far cadere separatezze, divisioni inutili nell'ambito giudiziario. Qui si chiede un parere al Consiglio superiore della magistratura come per altro aspetto abbiamo voluto che gli avvocati entrassero nei consigli giudiziari. Noi abbiamo voluto quell'inserimento perché riteniamo che sia corretto. Quindi la presenza del Consiglio superiore della magistratura, per la parte di sua competenza, non è e non deve essere una ingerenza. Gli avvocati, soprattutto di un certo livello, dovrebbero ragionare in maniera più serena e vedere nella presenza del Consiglio superiore della magistratura qualcosa in più, un *quid pluris*, qualcosa che qualifica sempre di più la figura e il ruolo dell'avvocatura, perché l'avvocato è un momento essenziale dell'amministrazione della giustizia e non può arroccarsi, in questo momento, come categoria, in una posizione culturalmente perdente. Quindi, quando noi chiediamo di sentire il Consiglio superiore della magistratura non vogliamo assolutamente togliere nulla all'avvocatura, semmai dare qualcosa in più.

contro questo emendamento, ma non ritengo né che mi si possa addebitare né una violazione del rispetto al massimo organo costituzionale che è il Consiglio superiore della magistratura... La manina così però no, senatore Maritati, perché l'hai detta grossa. Né tantomeno ritengo che i colleghi che sono contrari a questo emendamento si possano permettere il lusso di essere contro il Consiglio superiore della magistratura. Mai consentirò a nessuno di dire a me che sono contro il Consiglio superiore della magistratura.

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF. Non voglio entrare nella polemica che è stata già ampiamente e secondo me non correttamente portata avanti, perché qui non c'è proprio da fare polemica tra Consiglio superiore della magistratura, magistratura e avvocatura, ma si tratta di prendere atto che sostanzialmente si disciplina il praticantato presso gli uffici giudiziari saltando il parere del Consiglio superiore della magistratura sull'organizzazione dei corsi. Ciò è veramente incredibile e per questa ragione voterò contro l'emendamento 42.300 e chiedo il voto contrario del Gruppo.

Signora Presidente, io ero del tutto d'accordo con l'articolo 42 così come uscito dai lavori della Commissione,

molto ben tarato, di definire ulteriormente alcuni aspetti. Esso recita testualmente: «Al precipuo scopo di favorire lo snellimento burocratico sotteso alla frequentazione del praticante degli uffici giudiziari, in tale regolamento»

In quasi tutte le professioni è stata eliminata la prova di accesso mediante preselezione informatica; recentemente anche per il concorso notarile. Questa legge deve disciplinare una moderna professione forense in cui è il merito a dover prevalere e quindi anche al momento del concorso saranno i migliori a superare le selezioni se adeguatamente formati e messi nelle condizioni di farlo. A questo punto la contrazione del loro numero diventa qualcosa in eccesso rispetto alla legge. La legge deve ridisciplinare una professione forense una professione adeguata ai tempi, che veda l'avvocato protagonista in Italia, in Europa e anche nelle sedi internazionali. Porre questa barriera all'accesso significa fare un passo indietro e impedire a tanti giovani talenti di accedere alla professione, perché spesso il quiz è una delle prove

con l'emendamento 45.901 della Commissione, che sopprime l'articolo 45, si elimina la prova informatica. Quindi, esprimo parere favorevole

Onorevoli colleghi, vi era una richiesta e un accordo di vari Gruppi di terminare la seduta alle

Presidente, questa mattina, davanti al Ministero dell'economia e delle finanze sono scesi in piazza a manifestare i malati di SLA con i loro familiari, e noi con loro. Essi chiedono al Ministro misure adeguate per l'assistenza. Ho appreso però, con soddisfazione, che la delegazione dell'associazione dei malati è stata poi ricevuta dopo questo incontro, il Governo ha preso un impegno a presentare un emendamento alla legge di stabilità. le vicissitudini del Governo non debbano portare ulteriormente queste persone malate, ancora una volta, ad essere prese in giro.

la leggenda della genesi e della nascita delle mafie, cioè la storia di Osso, Mastrosso e Carcagnosso, i tre cavalieri spagnoli che, partendo da Toledo in Spagna, emigrarono nel Sud Italia dove fondarono la mafia in Sicilia, la 'ndrangheta in Calabria e la camorra in Campania. Fino a qui tutto bene. Sono notizie anche interessanti, che di sicuro attirano l'attenzione della gente. Però, poi, il monologo continua e lo scrittore conduttore televisivo cambia i soggetti della favola e li attualizza:

il centesimo candidato leader del centrosinistra. Noi della Lega Nord dobbiamo riconoscere con consapevolezza la grande bravura strategica, la diabolica perfidia di chi utilizza lo strumento televisivo, pagato tra l'altro con il canone di noi contribuenti, per colpire chi veramente, con i fatti e con i risultati, da oltre due anni combatte e mette in ginocchio il sistema mafioso nel nostro Paese: il ministro Maroni. mafiosi arrestati in due anni, il 50 per cento in più rispetto al Governo precedente. Altro che favole! Altro che i cavalieri Osso, Mastrosso e Carcagnosso.

Signora Presidente, il Ministro dell'interno, di cui cui parlavano i colleghi della Lega Nord, dal 20 aprile 2009 non risponde a numerose interrogazioni. Una di queste è indicata con il numero Il problema, signora Presidente, è che questa interrogazione riguarda dipendenti delle forze dell'ordine ora in trattamento in quiescenza, che hanno servito lo Stato per meriti particolari e che si trovano ora ad essere sfrattati dagli alloggi di servizio, dallo Stato a loro concessi mentre prestavano servizio in favore nostro e delle nostre istituzioni.

e credo che una sollecitazione possa essere rivolta al Gabinetto del Ministro dalla Presidenza del Senato, affinché la delicatezza e l'importanza della situazione siano sottoposte al ministro Maroni, così attento a molte altre realtà, in modo tale da poter rispondere con dovizia di particolari a una questione di cotale gravità.

si è verificata una situazione davvero complessa e singolare: due assessori regionali in carica sono stati raggiunti da provvedimenti giudiziari. Uno di essi si è dimesso; l'altro, l'assessore alla sanità (peraltro in una Regione nella quale questo settore importantissimo è stato commissariato in quanto soggetto al piano di rientro) è stato raggiunto prima da un provvedimento di restrizione, di arresti domiciliari, e successivamente da una misura più attenuata, da un provvedimento di obbligo di dimora. In sostanza egli non può muoversi dalla sua città e, quindi, non può partecipare alle riunioni della Giunta.

di una situazione istituzionale gravissima e questa circostanza da ieri si è ulteriormente aggravata. Questa è la ragione per la quale sollecito davvero con urgenza una risposta alla mia interrogazione.

si sta verificando una situazione al limite della violazione di principi costituzionali relativi al funzionamento dell'organo collegiale di governo della Regione Abruzzo. Per questo - ripeto - sollecito vivamente il Ministro dell'interno a riferire in Aula su che cosa sta accadendo in quella nostra, cara, martoriata regione. Presidente, sento il dovere di intervenire per associarmi a quanto detto dalla senatrice Biondelli e per informare l'Assemblea che i malati di sclerosi

Presidente, intervengo per sollecitare la Presidenza del Senato, pur nella contingenza dell'attuale situazione politica, a calendarizzare il

alle definizioni più aggiornate dell'Organizzazione mondiale della sanità. Rispetto a tutto ciò, l'intervento dello Stato, l'iniziativa del Governo,

riguarda i diritti negati al lavoro e all'assistenza.